qualche ora fa le agenzie hanno battuto la notizia di una nuova strage di civili a Gaza. A Beit Hanun sono stati uccisi nel sonno almeno diciotto palestinesi da un bombardamento indiscriminato delle forze israeliane, che ieri invece si erano ritirate dai Territori. Oggi dobbiamo sottolineare la nostra ulteriore deplorazione e il nostro sgomento verso questa nuova strage di civili che troppo ci ricorda l'orribile strage di Cana di qualche mese fa nel corso della campagna di attacco militare al Libano; un attacco non soltanto a popolazioni civili inermi, ma anche al tentativo estremamente difficoltoso del Governo palestinese di creare un Governo di coalizione e di unità nazionale, perché interviene proprio nel momento in cui Hamas e Fatah stavano intrattenendo dei colloqui per cercare di risolvere la grave crisi di *impasse* e stallo che attraversa il Governo nei Territori. Oggi Hamas chiede la convocazione immediata del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, e questo ci sembra un messaggio importante perché riconosce la legittimità di un foro internazionale e del diritto internazionale come chiave di soluzione di questa secolare controversia. però un ostacolo al lavoro che anche il nostro Governo sta giustamente facendo per costruire un percorso per una conferenza internazionale di pace che riconosca il diritto di due Stati di coabitare in sicurezza.

sulle misure che intende intraprendere per condannare questo episodio e riattivare i canali negoziali per risolvere questa crisi. *(Applausi

esprimere dei giudizi apodittici se non sono sostenuti da fatti realmente accaduti. È certamente doloroso il fatto che siano coinvolti dei civili in un'operazione militare,

davvero in una situazione in cui si possa dire: uccisi dalla barbarie e sepolti dall'oblio. Da troppo tempo lo Stato di Israele si permette, contro tutte le leggi internazionali, azioni contro civili ed occupa territori che l'ONU gli ha già chiesto ripetutamente di lasciare dal 1967. Credo che il Governo debba venire a riferire in Aula in modo che, finalmente, anche noi si possa

giusto che il Governo venga a riferire e - io credo - non solo sulla situazione dei Territori palestinesi, ma anche, aggiornandoci, sulla situazione e sul processo di pace in Libano, dove sono migliaia di nostri soldati. Penso che questo sia un impegno che il Governo ha preso e che deve mantenere, per cui non si può considerare l'area soltanto parzialmente. Proprio perché chiediamo al Governo di riferire, credo non sia il caso di formulare giudizi completamente schierati da una sola parte, che non tengono conto degli attacchi che vengono da territori

Signor Presidente, devo chiedere a lei e all'Assemblea la possibilità di proseguire ancora per un'ora i lavori della Commissione.

potremmo utilizzare quest'ora e mezza in maniera proficua affrontando il provvedimento che abbiamo lasciato sospeso nella giornata di ieri,

potremmo almeno utilizzare quest'ora e mezza per completare la discussione generale. Ci sono ancora cinque, sei o sette interventi e credo che questo sarebbe utile a tutti anche per evitare

La volevo ricordare perché è stata senatrice, è stata anche deputata, ma ha rappresentato per le donne italiane - credo tutte le donne italiane - un punto di riferimento per molti anni. Fu sua l'idea della Commissione nazionale per le pari opportunità, il primo strumento di parità introdotto nel nostro ordinamento, che presiedette a partire dal 1984.

in quel Codice donna che è diventato una buona prassi in molti Paesi europei. Era un'amica delle donne, era un grande avvocato, era una socialista appassionata. Chi l'ha conosciuta ricorda certamente la sua passione, la sua capacità di interpretare in maniera autentica e sincera la politica e la sua grande passione politica. Ma credo che la ricorderanno anche per la sua solarità, per la sua capacità di essere amica delle donne in qualunque schieramento si trovassero e di essere appassionata ricercatrice degli strumenti, delle strade, delle parole che potessero aiutare le donne italiane ad occupare la scena pubblica della politica, dell'economia. È sua l'intuizione della legge sull'imprenditoria femminile, che ha aiutato moltissime donne italiane a far valere il proprio talento, la propria ambizione, la propria capacità di mettersi nel mondo imprenditoriale così ostico alla presenza femminile, superando la barriera del credito, così spesso precluso alle donne. Credo che non vi sia stata una sola occasione importante, in cui si ragionava di questo, nella quale Agata Alma Cappiello non fosse presente. Anche coloro i quali non l'hanno conosciuta direttamente credo la ricordino per questa semplice passione di stare nel mondo della politica, di stare dalla parte delle donne, di stare - lasciatemelo dire - anche dalla parte dei soggetti più deboli ed esposti, a valorizzare e riconoscere diritti. So che non è un argomento sul quale abbiamo tutti la stessa opinione, ma vorrei ricordare che vent'anni fa la prima proposta di legge in materia di riconoscimento delle coppie di fatto fu di Alma Cappiello. Di lei ho troppi ricordi personali per poter essere probabilmente pienamente ufficiale in questa commemorazione: troppo lavoro, troppe riunioni, troppi luoghi, troppe tappe vissute insieme. Mi pareva, però, giusto che il Senato la ricordasse per il suo lavoro, che ne ha fatto, in anni anche molto, molto difficili, per il suo partito (era una socialista, come sapete, limpida nella sua adesione convinta) una dirigente politica. Spesso queste parole vengono usate per gli uomini; io credo che ora vadano spese pienamente, con piena legittimità, per ringraziare Alma della sua generosità.

espresse, anche con particolare commozione, da parte della senatrice Finocchiaro per ricordare Alma Cappiello: come ha detto lei, una socialista vera,

dovere di ricordare queste caratteristiche che hanno costantemente informato la vita politica di Alma Cappiello perché sono stato nel Gruppo parlamentare socialista insieme a lei qui al Senato e debbo dire che Alma Cappiello, soprattutto nella legislatura che fu contraddistinta da quel ciclone giudiziario che fece scomparire la cosiddetta Prima Repubblica, era campione nella difesa di princìpi fondamentali della giustizia, quella vera, non quella giustizialista, e della libertà e democrazia. Purtroppo anche Alma Cappiello fu vittima di quel giustizialismo che fece *tabula rasa* di quei partiti che avevano garantito al nostro Paese libertà e democrazia. Mi piace quindi ricordarla proprio perché rappresentava un pilastro fondamentale, soprattutto al Senato, nel sostenere queste battaglie che rimangono irrinunciabili. Mi fa piacere anche che le considerazioni svolte dalla senatrice Finocchiaro vengano come espressione anche di un Partito che fece dell'aggressione giudiziaria una costante della politica, in Parlamento e fuori da esso. Alma Cappiello fu vittima di questa politica giustizialista, perché il Gruppo socialista, come ricordiamo, scomparve dalle Aule parlamentari in relazione all'aggressione che si consumò, in modo direi disgraziato, nel nel nostro Paese. Non voglio oggi continuare a riaprire ferite o polemiche di questo tipo, però credo che, nel momento in cui ricordiamo una grande socialista autonomista, democratica, riformista, profondamente legata ai valori della libertà e della democrazia,

iniziativa e la continuità nella sua vita parlamentare proprio a causa degli attacchi dell'azione giustizialista che fu portata avanti con determinazione nel nostro Paese con l'idea e l'obiettivo di distruggere la tradizione socialista (che, guarda caso, oggi viene costantemente ripresa), nonché le

Propongo un attimo di raccoglimento a ricordo della nostra ex collega.

con una serie di audizioni e con una missione in Campania che ha consentito di portare a conoscenza della Commissione una situazione di una gravità estrema. La Regione Campania si in emergenza dal febbraio del 1994, quando fu dichiarato appunto lo stato di emergenza e fu nominato un commissario per l'emergenza rifiuti in quella Regione. In quell'anno il problema dei rifiuti era legato soprattutto era legato soprattutto all'emergenza criminalità, perché le discariche erano gestite in gran parte dalle organizzazioni criminali di tale Regione.

il commissariamento al presidente della Regione Campania, e così è stato dal 1996 fino al 2004, con il succedersi di tre presidenti della Regione Campania con poteri commissariali: i presidenti Rastrelli, Losco

dopo le dimissioni dello stesso e con l'esplodere dell'ennesima emergenza rifiuti nella Regione Campania, il Governo interviene ancora con un decreto per nominare commissario straordinario il Capo del Dipartimento della protezione civile. Già tale scelta ci dà il senso della drammaticità della situazione che la Regione Campania sta vivendo in questi mesi.

sia facile per ognuno di noi fare un'analisi critica di ciò che è avvenuto in questi anni. Ricordo a me stesso e a tutti i colleghi che in dodici anni si sono succedute amministrazioni e Governi regionali di centro-destra e di centro-sinistra e Governi nazionali di centro-destra e centro-sinistra e purtroppo la situazione non è cambiata. Oggi nella Regione Campania abbiamo circa 40.000 tonnellate di rifiuti sparse per le strade, più 7.200 tonnellate che vengono prodotte ogni giorno e rispetto alle quali non c'è soluzione, non ci sono impianti. Era stato predisposto un fu fatta un gara, annullata anche con questo ultimo decreto; non abbiamo ancora gli impianti che completano l'intero ciclo, la filiera del ciclo dei rifiuti. Quindi,

prevista in un decreto - quello alla nostra attenzione per la conversione - della riapertura delle discariche. Ci sono dei numeri che credo servano a tutti i colleghi per comprendere perché siamo alla più grave crisi di emergenza in tale Regione.

ingente quantità di rifiuti a impianti di incenerimento o a discariche occorrerebbero dei decenni. I calcoli che sono stati fatti in Commissione bicamerale nella passata legislatura ci indicano dai 35 ai 50 anni per poter smaltire il carico di rifiuti accumulati negli anni passati in Regione Campania. Campania. Ci sono sicuramente delle gravi responsabilità, sulle quali non credo che si possa più tacere, ma sono responsabilità lunghe dodici anni, che segnano un'incapacità gestionale di programmazione e di elaborazione di un piano capace di rendere quella Regione in grado di poter - analogamente a quanto avviene in altre parti del Paese - segnare un punto di svolta e di uscita definitiva dall'emergenza.

senza alcun piano regionale e senza l'indicazione da parte dell'organo regionale dell'individuazione dei siti, gli impianti. Si stabilì con quella gara nata nel 1996, formalizzata nel 1998, conclusa nel 2000, quindi attraverso Rastrelli, Losco e Bassolino, commissari all'epoca, che a decidere dove costruire gli impianti sarebbe stato un soggetto privato e non pubblico, venendo meno a qualsiasi logica

del San Marzano doc, quella di Acerra. Da ciò nascono proteste, mobilitazioni, che portano all'apertura di un cantiere ad Acerra con un dispiegamento di forze dell'ordine e grandi sommovimenti popolari, mentre il cantiere di Santa Maria La Fossa ancora oggi

appunto con un pagamento a piè di lista, fior di quattrini (85 milioni di euro in dieci mesi). E per che cosa? Per gli impianti, per i siti di stoccaggio. Qui

con il meccanismo delle ordinanze commissariali e spesso con le ordinanze della Presidenza del Consiglio dei ministri, si sono fatte molte storture, si sono avallate molte operazioni ai limiti della legalità; alcune delle realtà che citavo sono frutto di ordinanze commissariali che, in deroga a qualsiasi normativa, forzavano per aprire lo spazio, o comunque non chiudevano le porte alle organizzazioni criminali. L'articolo 2 è importante: in esso si riconosce il senso dell'informazione e della partecipazione dei cittadini

contro la volontà delle comunità, degli enti locali, ma vanno fatte di concerto con le amministrazioni, con le comunità, in un processo partecipato che consenta di avere scelte condivise che non dovrebbero determinare le tensioni e i conflitti che si sono avuti negli anni passati. L'articolo 3 tratta dell'affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti, attribuendo al commissario la facoltà di intervenire con somma urgenza (quindi, anche qui in deroga, anche con la possibilità della trattativa privata, per cui credo che sia maggiormente importante porre limiti temporali rispetto a questa azione) per individuare i soggetti che possano

(CDR o non CDR, come vogliamo definirlo), questa montagna di rifiuti che abbiamo in Campania, per poterla anche avviare verso le cave dismesse e abbandonate, una volta messe in sicurezza.

scivolare nella polemica politica. Il tema è particolarmente delicato, per cui invito, come è avvenuto in Commissione, tutti i colleghi a fare uno sforzo per comprendere che questa deve essere l'ultima volta che il Parlamento si occupa di una Regione, della Regione Campania, del tema dei rifiuti. Vorrei che il Parlamento si interessasse di altro, magari dei rifiuti, ma rispetto a un piano nazionale per portare il nostro Paese verso gli obiettivi che altri Paesi europei si sono dati in tema di ciclo dei rifiuti. Purtroppo, siamo costretti ad occuparci di questa situazione, questa situazione, che è talmente drammatica che non può che essere affrontata anche con l'intervento del Governo centrale, appunto con l'auspicio che sia l'ultima volta. *(Applausi dai

di un problema ormai assolutamente irrisolto e credo irrisolvibile anche alla luce del decreto-legge che è oggi al nostro esame. Vorrei ricordare ai colleghi che negli ultimi 12 anni per il problema dell'emergenza perenne dei rifiuti in Campania

non dei Comuni, non della Regione, non delle Province della Campania: un miliardo e mezzo proveniente dalle tasche di tutti quei cittadini che pagano normalmente le tasse. poi del pagamento delle tasse, vorrei rinfrescare la memoria sul peso tributario che grava in modo assolutamente diverso nelle varie latitudini della nostra Nazione. infatti, a Napoli la pressione tributaria è di circa 400 euro *pro capite*, a Milano è di circa 700 euro *pro capite*.

Ancora una volta, però, si ricorre a misure forzose per risolvere il problema, mai neanche affrontato, della costruzione di termovalorizzatori, che i cittadini campani sono bravissimi bravissimi a contrastare. I cittadini campani sono bravi a portare le carrozzine con i bambini sui binari della ferrovia, in 2.000, 3.000; addirittura i sindaci, non più tardi di due settimane fa, hanno bloccato una ferrovia. È una cosa inaudita in questa Nazione, se solo si ricordano i blocchi fatti dai Cobas! Signori, lo ripeto, bisogna trovare il sistema di far pagare chi ha sbagliato, anche penalmente, perché, come ho già detto (ma lo ripeto), gli amministratori campani o sono ladri o sono incompetenti.

I Presidenti delle Regioni devono essere d'accordo, non basta ascoltarli, signor Presidente. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio innanzitutto il relatore per aver sottolineato il clima del dibattito e del confronto all'interno della Commissione. Abbiamo affrontato un problema delicato nella consapevolezza di essere una forza politica che ha avuto responsabilità di Governo e che, nel momento in cui è chiamata a svolgere un ruolo di opposizione, non può dismettere la cultura istituzionale e la cultura di Governo. Lo abbiamo fatto con grande senso di responsabilità, ma anche con grande chiarezza e determinazione; chiarezza e quella determinazione che ci impongono di evidenziare un *vulnus* determinante di questo decreto-legge, prima ancora che nell'articolazione della proposta di merito nell'impostazione di carattere finanziario. Allo stato, si tratta di un provvedimento sostanzialmente privo di copertura finanziaria certa e reale. il meccanismo individuato rinvia a successivi aumenti tariffari, o meglio ancora a una presunta tassa regionale sui rifiuti solidi urbani. Ciò determina uno strano meccanismo per cui, rispetto ad un impianto che prevede una serie di poteri commissariali, si ottiene il risultato della tassa o della tariffa a piè di lista, vale a dire a copertura degli interventi e delle iniziative significative e notevoli che il commissario dovrà concretizzare per tentare di superare l'emergenza rifiuti. È una questione contabile ed insieme politica, perché significa scaricare le responsabilità dell'incapacità di governo sui cittadini della Campania attraverso inasprimenti di tasse e di tariffe, peraltro non predeterminabili in via preventiva, ma soltanto a seguito delle risorse che il commissario spenderà nella sua attività. Ebbene, credo che il primo punto sia questo: siamo disponibili a continuare un confronto responsabile, ma chiediamo innanzitutto alla maggioranza e al Governo di affrontare diversamente il tema della copertura finanziaria, che è una questione centrale non solo dal punto di vista contabile ma, lo ripeto e sottolineo, anche politico. Dico ciò anche in relazione all'intervento che mi ha preceduto poiché il problema che stiamo affrontando richiama alla dignità della politica e alla responsabilità delle istituzioni. Non è possibile continuare con il commissariamento: significa commissariare pezzi di sovranità e di rappresentanza popolare e deresponsabilizzare il ceto politico e istituzionale in Campania. Credo che chiunque abbia a cuore la dignità della politica debba porsi responsabilmente il problema del superamento del commissariamento e del ritorno a poteri normali. Mi chiedo, rivolgendomi anche all'intelligenza e alla sensibilità di quest'Aula, come sia possibile immaginare un Governo del territorio in Regioni dove ci sono il commissariamento dei rifiuti, il commissariamento per l'assetto idrogeologico, in sostanza tutta una serie di commissariamenti che gridano vendetta e che devono essere assolutamente superati. se consideriamo il dibattito politico che si svolge oggi, dopo che il centro-sinistra e la maggioranza hanno determinato nel Paese, prima, durante e dopo la campagna elettorale, l'utilizzo della centralità del Mezzogiorno come la grande metafora del cambiamento. Quella grande metafora che non si è tradotta nel documento finanziario

si determina un meccanismo perverso che penalizza i cittadini della Campania. In una Regione dove il sistema produttivo è chiamato, attraverso la maggiorazione dell'IRAP, a pagare l'ingovernabilità della sanità in Campania, si aggiunge una ulteriore tassa a carico dei cittadini, che devono pagare il malgoverno rispetto alla capacità di gestire i rifiuti nel territorio. Invito la maggioranza a riflettere su tutto questo. Come opposizione avremmo tutto l'interesse a cavalcare la propaganda anziché affrontare e risolvere i problemi. invece, che la politica si misuri attraverso la capacità di affrontare i nodi: non cavalcarli, ma affrontarli. Siamo pronti ancora una volta, lo ribadisco, ad affrontare questo tema con grande senso di responsabilità, ma individuando il superamento di un meccanismo di copertura che è inaccettabile. Prima ancora di intervenire nel merito e quindi nel dibattito sugli emendamenti, chiedo che si svolga una riflessione preliminare su questo punto, che è fondamentale ai fini della prosecuzione dell'intervento e del dibattito. Questa è la nostra posizione. Tra l'altro vorrei ricordare un aspetto, avviandomi alla conclusione. Signor Presidente, il dato paradossale è che mentre si prevede l'inasprimento della tassa a piè di lista, con questa sorta di finanza di progetto applicata ai rifiuti, a tariffa, sostanzialmente - in un modo che è anche esplicitazione di una capacità creativa di fare finanza - nello stesso tempo, rispetto al disastro ambientale e al problema della tutela della salute derivante da quella straordinaria ed ignobile vicenda dei rifiuti in Campania, si dimentica che ancora oggi

il servizio abbiano la possibilità di attivare meccanismi tali da consentire la detrazione della tassa che pagano per un servizio che non ricevono. ricevono. Ciò è previsto dal comma 6 dell'articolo, che consentirebbe tale esercizio legittimo da parte dei cittadini che non trovano risposta. Il Governo e la maggioranza,

e il senso di responsabilità che dobbiamo avere rispetto allo sviluppo di quella terra dalla straordinaria potenzialità e anche dalla straordinaria positività. In Campania e nel Mezzogiorno, infatti, non vi è soltanto il cumulo dei rifiuti, ma vi è anche un grande cumulo di intelligenza, di energia, di positività,

e recuperiamo il dibattito che abbiamo svolto in Commissione, in cui abbiamo posto un termine a questa vicenda: entro il 2007, se non prima, bisogna chiudere il commissariamento, tornare alla gestione dei sindaci, dei preti, dei Presidenti di Regione, i quali si devono assumere le responsabilità. Il vero modo per rispondere a coloro i quali, su tutti i grandi giornali e quotidiani, oggi parlano in un certo modo della Campania non è l'isterismo di chi governa le istituzioni,

con i commissariamenti, ritorniamo alla dignità della politica e alla qualità delle istituzioni.

signor Sottosegretario, colleghi senatori, penso che quella fornita al Governo e al Parlamento dalle dimissioni del prefetto Catenacci, quale commissario delegato per l'emergenza rifiuti, sia, in ordine temporale (e per questo ritengo anche più colpevole), l'occasione sprecata, attraverso il decreto-legge che siamo chiamati oggi a convertire in

è mancato il coraggio, considerata anche la fase difficile che vive la Campania in materia di rifiuti, che qualcuno ha giustamente definito di "emergenza nell'emergenza". Atteso quindi anche questo momento difficile, noi riteniamo che al Governo sia mancato il coraggio per indicare, nel decreto-legge, una via di uscita dalla fase della gestione straordinaria di tipo commissariale: non c'è una indicazione, un percorso, una soluzione ponte che porti la gestione straordinaria a quella ordinaria. Sono passati dodici anni e ci avviamo verso il tredicesimo anno. L'11 febbraio del 1994 fu la data del primo commissariamento della Regione Campania per affrontare l'emergenza rifiuti.

tipizzate come rifiuti nobili da poter convertire in energia elettrica, in realtà forse sono qualcosa di molto vicino al rifiuto solido da sversare in discarica. Nulla è cambiato rispetto al 1994 nemmeno per quello che riguarda le politiche di smaltimento. Politica della discarica, quella portata avanti nella prima emergenza nel 1994,

politiche della discarica ancora oggi, perché questa è l'unica politica possibile, visto il fallimento di tutti i programmi integrati per smaltire il rifiuto attraverso un ciclo completo. Da ultimo, basta richiamare il fallimentare piano adottato dalla gestione commissariale Bassolino, presidente della Regione Campania e commissario, in data 30 settembre 2002. Tutto come nel 1994, salvo la realizzazione, nel frattempo, di sette impianti per la produzione del cosiddetto CDR (combustibile da rifiuto)

realizzati per la protesta delle popolazioni, nonché per qualcos'altro che tutti conosciamo, ma che non si affronta con le dovute energie. Né penso che il fallimento del piano sia da addebitare esclusivamente alla sfasatura temporale fra la realizzazione degli impianti per la produzione del CDR e i termovalorizzatori. PRESIDENTE. Senatore Morra,

che afferiscono a questo piano. Bene, tutto ciò doveva suggerire a questo Governo un maggior coraggio perché noi pensiamo, al di là

dal Governo e dal Parlamento; un po' da tutti i Governi e in misura maggiore da questo perché è l'ultimo in ordine temporale. Il tutto è avvenuto per un cattivo uso, per un abuso - direi - distorto dello strumento del commissariamento.

delle Province e dei Comuni. Attraverso questa deresponsabilizzazione si è infilata la mafia, la camorra, il malaffare.

Vorrei dire soltanto che non si può invocare - come fa questo decreto - la solidarietà nazionale in un contesto territoriale, quale quello campano, completamente deresponsabilizzato, Concluda, non mi costringa a toglierle la parola.

Nella relazione, il collega Sodano accennava ad alcuni dati che devono essere oggetto della nostra riflessione. Ci troviamo di fronte ad un commissariamento che ormai perdura nel tempo,

Questa situazione drammatica ha delle responsabilità. Mi spiace doverlo sottolineare, ma credo che l'Aula non possa fare a meno di sottolinearle. Sono responsabilità che, per la verità, non possono essere - com'è noto - scaricate da una parte o dall'altra, ma responsabilità che credo la classe politica che ha governato negli ultimi tredici anni

cause delle gravi crisi che si sono succedute nel tempo fino ad oggi è da rintracciarsi proprio nell'aver

danni non solo ambientali, ma anche economici molto forti alla Regione. Penso ad alcune zone, tra l'altro di agricoltura di qualità, che hanno già tanti problemi per le varie discariche

I commissariamenti che si sono succeduti in questi anni hanno operato sulla base di un vecchissimo piano dei rifiuti; non hanno fatto praticamente nulla per la raccolta differenziata, né per

Deve essere l'ultima volta e ognuno si dovrà assumere le proprie responsabilità fino in fondo per fare in modo che si esca una volta per tutte dall'emergenza...

un incontro a Napoli sulla questione della sicurezza e sempre in relazione alla Campania oggi ci troviamo a dover discutere dell'emergenza infinita relativa allo smaltimento dei rifiuti. Per noi è significativo il modo in in cui il Governo affronta la questione: non incarica una figura qualsiasi, bensì il Capo del Dipartimento della Protezione civile nazionale, incernierato sulla Presidenza del Consiglio dei ministri. La Protezione civile nazionale, colleghi, interviene nei momenti di emergenze nazionali: dissesti idrogeologici, disastri immani, catastrofi. Questo sta a significare che il nostro Governo ha classificato come catastrofe di valenza nazionale l'incapacità di gestire una delle attività più banali, che è un servizio pubblico a carattere comunale, e cioè mettere da una parte e smaltire i rifiuti che si producono quotidianamente: non un avvenimento straordinario ed eccezionale, ma l'ordinarietà che tutte le amministrazioni comunali devono fronteggiare quotidianamente. Come la fronteggia questo Governo? Probabilmente nel modo italiota, cioè nel modo in cui non si vogliono mai risolvere le questioni: si nomina un commissario - «speciale», a questo punto - ma lo si pone nella condizione di avvalersi di una sub-burocrazia inventata per decreto, cioè altri tre subcommissari. Scusate, forse conosciamo poco la struttura amministrativa della Campania, ma esistono uffici, direzioni generali, esistono funzionari e direttori generali, anche in parte responsabili, i quali avrebbero dovuto obbligatoriamente affiancare il commissario! Secondo il sistema italiano, si crea invece burocrazia su burocrazia: si affiancano nuovi tre subcommissari e, addirittura, il commissario delegato potrà nominarsi una commissione di esperti. Quando sentiamo queste premesse, pensiamo subito: «e i costi»? Ebbene, probabilmente anche il Governo si è posto questa domanda e infatti afferma che i costi non dovranno superare i preventivi o comunque l'ordinario, nel senso che i maggiori oneri dovranno essere affrontati con riduzione di personale presso le strutture commissariali. Signore Iddio, peggio di così non è possibile! Riduciamo personale operativo e nominiamo capi. Ma voi pensate che solo a livello dirigenziale si risolvano le questioni? *Todos caballeros*. Un esercito di generali. Ma cosa farà operativamente?

le procedure di gara iniziate - e può essere che sia una buona cosa - e affidare in modo diretto tutte le attività le attività che servono per affrontare l'emergenza. Sappiamo cosa significa: affidamenti diretti, procedure *extra legem*, extra evidenza pubblica: che poteri si vanno a concentrare sul commissario!

scrivere nel decreto che il commissario avrebbe potuto stabilire di trasferire rifiuti anche in altre Regioni, semplicemente previa consultazione con gli altri presidenti, significava commissariare tutti gli altri presidenti regionali e superare l'autorità

l'UDC è stata contraria al commissariamento fin dal primo momento, anche se è consapevole del problema che esiste in Campania.

presidente, che non si degna di ascoltare il Parlamento e una sua Commissione, che non è responsabile insieme al Senato di questo grave problema ma che con grande senso di responsabilità e consapevolezza intende lavorare

perché questo territorio è massacrato dai rifiuti. In Campania è umiliata la dignità dei cittadini, che in certe realtà e momenti si sono trovati nell'impossibilità di andare la domenica a messa o di mandare i ragazzi a scuola. Penso sia un fatto veramente grave e mai a sufficienza evidenziato. Ho detto che si tratta di un problema nazionale: è infatti un problema nazionale quello dei rifiuti, che è molto più forte in Campania. Qualcuno ha detto in Campania ogni volta che si decide di fare qualcosa, c'è la ribellione. È vero, ma questa ribellione c'è anche da altre parti perché non dimentichiamoci quello che è successo a Venaus con la TAV: la gente scende in strada e blocca le opere pubbliche. cosa manca? Molte volte manca una classe politica che abbia la capacità di guidare e di assumersi delle responsabilità, quello che è successo in tutti questi anni in Campania. In Campania sono stati spesi tanti soldi - è stato detto prima - dei cittadini italiani. Un Parlamento ha il dovere di operare con senso di giustizia e tengo a ricordare - non dimentichiamolo - che in Campania c'è tanta gente onesta che ogni giorno lavora e paga le tasse, paga la tassa sui rifiuti e si trova i rifiuti per strada; paga una tassa per un servizio che non le viene dato. E gli amministratori cosa fanno? Non ne rispondono, non sono capaci di dare un segnale forte al cambiamento in quest'area del Paese e, dico io, in tutto il Paese. i dati di allarme del prefetto di Napoli sulla questione della criminalità legata al problema dei rifiuti, i dati allarmanti del commissario Catenacci, il problema dei contratti, il problema della gestione economica dell'emergenza e - ciò che mi preoccupa di più - i dati allarmanti di Bertolaso, che è venuto in Commissione il primo giorno a dire che avrebbe risolto il problema emergenza in dieci giorni. Mi sono permesso di avere dei dubbi ma voglio ma voglio ribadire la nostra stima e il nostro rispetto per il commissario Bertolaso. È proprio per questo che all'inizio ho detto che abbiamo molti dubbi sul commissariamento, perché si rischia di lasciare questo commissario da solo a risolvere un problema che, bene o male, non è il suo, o non è solo il suo, o è il suo in minima parte. Dicevo che gli amministratori locali, alla richiesta di informazioni, si permettono di essere latitanti e di non rispondere. Il 40 per cento dei Comuni non risponde alle richieste informative da parte dei prefetti; sono dati allarmanti sui quali il Parlamento, secondo me, dovrebbe veramente riflettere. Ricordiamoci che il commissario Bertolaso ha detto che ha paura di lottare contro i mulini a vento a vento e che ha paura di lavorare con chi non ha la voglia di risolvere questo problema (è agli atti della Commissione). un altro problema grave da considerare. Come ho già detto, in Campania ci sono, come in tutte le Regioni, forse in misura maggiore, cittadini disonesti ma anche tanti cittadini onesti che pagano le tasse. E qual è la soluzione per l'emergenza rifiuti che ci dà questo decreto? Quella di scaricare sulla tariffa i costi dell'emergenza. Scaricare sulla tariffa vuol dire far pagare non a chi evade le tasse ma a chi la tassa sui rifiuti paga un servizio per il quale ha già pagato, un servizio

in Commissione, maggioranza e minoranza si sono trovate spesso d'accordo nel valutare l'inconsistenza, o il problema per cui questo decreto rischia molte volte di non stare in piedi. Faccio un esempio un esempio che riguarda la storia dei rifiuti: il problema della FIBE. È già stato detto, ed è un assurdo, che da quando è stato rescisso il contratto, la FIBE incassa molto più di prima. Possiamo dire che quasi incassa *cash* il pagamento dei servizi effettuati: un fatturato, negli ultimi dieci mesi, di 85 milioni che sicuramente è già stato pagato per 50 milioni di euro, ma c'è chi sostiene che sia già stato pagato in questi giorni fino a 80 milioni. Nessuna società che lavora per lo Stato o per un ente pubblico riesce ad incassare i propri proventi in tempi così rapidi. Nel concludere questo mio intervento, voglio ricordare ancora i problemi economici. Dobbiamo - e speriamo che nel corso di questo dibattito si possa farlo - trovare una soluzione vera, che non è quella di scaricare sui cittadini campani i costi. Ricordiamo che il commissario ha detto che il *deficit* è di 5 milioni di euro al mese; sono tra i 12 e i 16 milioni di euro al mese le spese e i costi per la gestione dell'emergenza. Come recuperiamo tali costi? Il Governo ce lo deve dire; non può lasciare

loro operato la Commissione di merito e il presidente Sodano, che ha lavorato con grande capacità e con senso di responsabilità. Mi associo al suo auspicio: deve essere l'ultima volta che il Parlamento si occupa di questi problemi. Sono problemi degli enti locali, del governatore - ma preferisco chiamarlo presidente Bassolino, dei sindaci e dei Presidenti che non partecipano a questa emergenza. Speriamo che i cittadini se ne accorgano. La politica dei rifiuti devono farla gli enti locali.

ricordare all'Aula che ieri abbiamo comunicato che in chiusura procederemo al voto segreto sulla reiterazione

è evidente che la conversione in legge di un decreto, che ha come oggetto misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti, parte da un dato oggettivo che ha illustrato molto bene il relatore, presidente Sodano: l'emergenza c'è. Sicché, francamente, qualche battuta sul tema, che sarebbe stato meglio un ruolo diretto delle istituzioni o una maggiore programmazione, bisogna evitarla come battuta superficiale, se non si va - come bene ha fatto il senatore Sodano - a ricostruire la storia

da quando fu varato il vecchio piano - per pura cronaca, fu varato dall'allora presidente della Giunta regionale, senatore Rastrelli - è un dato che quel piano, portato avanti certamente anche dalla successiva Giunta di Bassolino, non ha funzionato e un gestore - ne ha parlato il collega che mi ha preceduto - quale la FIBE (che non è una società locale napoletana, ma l'unione di grandi gruppi italiani e stranieri, il cui protagonista si chiama Impregilo) ha lavorato malissimo, con sospetti che non io, ma la Commissione d'inchiesta nella passata legislatura ha evidenziato, creando un'emergenza sanitaria, ambientale e di ordine pubblico. Non facciamo allora facili demagogie sull'ordinario che noi vogliamo, insieme ad altri e più di altri, come parte politica, sul ruolo degli enti locali e sulla programmazione del ciclo dei rifiuti. Anch'io mi associo al ringraziamento a tutta la Commissione ambiente del Senato, maggioranza e opposizione, per il buon lavoro svolto e permettetemi di ringraziare il presidente, senatore Sodano.

che rischia di perpetrare un'altra gara ambigua di cui ancora paghiamo gli effetti e la delega al commissario a individuare soluzioni idonee per lo smaltimento dei rifiuti e delle ecoballe, anche eventualmente con affidamenti diretti sottolineo - a società diverse da quelle oggi attive e che gestiscono il servizio. La seconda novità è la grande attenzione alla raccolta differenziata che -aggiungo - la Commissione,

strane polemiche, seppur giuste, sul fatto che poi, alla fine, sono i cittadini a pagare anche l'aumento dei costi causati da una cattiva gestione. Non v'è dubbio che, in riferimento alla Carta di Aalborg, l'informazione e la partecipazione siano il principale antidoto ai rischi evidenziati. l'utilizzo della struttura operativa nazionale della protezione civile. Anche qui, rispetto agli altri commissariamenti (prima ai Presidenti delle Regioni, poi al prefetto Catenacci), questa sinergia tra struttura commissariale e nazionale dalla protezione civile, a nostro avviso, è importante, anche nel sottolineato rapporto con gli enti locali con la Regione, per definire i piani della raccolta differenziata e - perché non dirlo - per avviare la preparazione da parte degli enti locali e della Regione di un nuovo piano. il primo obiettivo cui, come forza politica, lavoreremo a livello nazionale e locale. Perciò, anche il monitoraggio previsto dal decreto e la commissione di esperti sono fatti utili. Il tutto - voglio ricordarlo - con invarianza di spesa,

non capiremmo questa storia, in cui - sia chiaro - sicuramente tutte le parti politiche, anche chi governa attualmente la Regione e i Comuni

sul ciclo integrato, sulla trasferenza, sulla termodistruzione e sulla raccolta differenziata. Non capiremmo la situazione attuale se non vedessimo qual era quella precedente. In secondo luogo, oltre a parlare dei limiti della Regione, della Provincia e dei Comuni, guardiamo - come ho già ricordato - alla responsabilità della FIBE e, soprattutto, poniamoci il problema di com'è stato possibile pensare che un privato potesse individuare i siti e costruire gli impianti, senza nessun rapporto con la programmazione e con i cittadini. credo che la relazione del senatore Sodano abbia messo in evidenza un aspetto importante, cioè la raccolta differenziata, rispetto al quale vanno sicuramente individuati strumenti e misure

del commissario Bertolaso, soprattutto per la citata esigenza di coinvolgere le strutture operative nazionali della protezione civile. Esprimiamo fiducia che questo Parlamento riesca a monitorare e a vigilare, affinché, nel tempo previsto da quest'ultimo commissariamento, enti locali, Regione e tecnici giungano a porre le condizioni di una nuova responsabilità delle popolazioni meridionali nella risoluzione di questo problema.

la parola. E' stato ricordato come noi del centro-destra abbiamo affrontato l'esame di questo provvedimento con grande senso di responsabilità, per cercare di dare soluzione ad una questione che riteniamo spinosa; tuttavia, non possiamo sostenere un provvedimento che, secondo noi, ancora aperti diversi nodi e non risolve il problema dell'emergenza. Molti di noi che veniamo dalla passata legislatura sappiamo bene che il Governo Berlusconi per ben due volte si è occupato della Campania e lo ha fatto con quella correttezza istituzionale che coinvolgeva gli enti territoriali, segnatamente la Regione. Abbiamo l'impressione che con questo provvedimento il Governo abbia scaricato la Regione Campania, abbandonando i cittadini - lo voglio ricordare: sei milioni di cittadini - al loro destino sulla vicenda dei rifiuti. Tale vicenda - voglio rispondere al collega Sodano - ha delle responsabilità precise:

nel dirlo e, in proposito, vorrei invitare i colleghi a leggere la relazione conclusiva

a quest'Aula le dichiarazioni rilasciate alla stampa dal commissario Bertolaso e quello che ha detto a noi in una recente missione a Napoli. Bertolaso ha affermato: la mia è una battaglia contro i mulini a vento. Non riesco a trovare interlocutori, anzi vi è uno scaricabarile nei confronti del Commissariato. Ho l'impressione che qui in Campania non vi sia la volontà di risolvere il problema. Siamo profondamente preoccupati per la situazione che si è creata in Campania. Sottoscrivo in pieno quanto dichiarato

alla quale dovevano aderire i Presidenti delle Province e il Presidente della Regione per individuare i siti, abbiamo creato lo

sulle dimissioni presentate dalla senatrice Magnolfi. I senatori favorevoli ad accogliere le dimissioni premeranno il tasto verde al centro della postazione di voto; i senatori contrari premeranno il tasto rosso a destra; i senatori che intendono astenersi premeranno il tasto bianco a sinistra. Poiché si tratta di uno scrutinio segreto, qualunque sia la scelta di voto effettuata, la luce che si accenderà sarà di colore neutro. Dichiaro aperta la votazione.